è la rappresentazione distorta che i mezzi di comunicazione di massa forniscono delle donne. Anche questa è un'anomalia tutta nostra in Europa. È un'anomalia se le donne devono scendere in piazza per gridare il rispetto della loro dignità; ed è un segno di questa anomalia persino il fatto che il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio per l'8 marzo, abbia dovuto ammonire a non dare un'immagine consumistica delle donne,

prima mozione, signora Presidente, scritta circa tre anni fa, parliamo di immagine stereotipata offerta dai *media*, ma ora siamo ben oltre gli stereotipi. Lo abbiamo toccato con mano, leggendo i numerosi interventi da parte maschile alla vigilia delle manifestazioni del 13 febbraio: febbraio: in molti di quegli articoli si parlava della legittimità, quasi, dello scambio sessuale, presentato come libertà. No, colleghi. In quei ragionamenti c'è solo l'equivoco della libertà femminile. In realtà, si tratta di una forma aggiornata di assoggettamento del corpo delle donne ai voleri e ai desideri maschili. È una forma più insidiosa di sudditanza, travestita da libertà. Non c'è dubbio che il modello televisivo di donna leggera, che sta nuda e muta sulla scena, bella e zitta, è enormemente pervasivo, penetra nelle coscienze di tante giovani donne, di adolescenti, e le condiziona. È il modello del successo facile, ottenuto attraverso l'esibizione del corpo, del diventare famose a tutti i costi, anche a costo di prostituirsi. Poco arriva sui *media* della realtà normale di donne che faticano per affermarsi perché sono brave, istruite e capaci. Del modello rappresentato da queste donne che raggiungono traguardi importanti per le loro capacità nelle professioni, nella ricerca, nell'imprenditoria, nella politica, nell'associazionismo, nelle istituzioni, nell'arte e nella cultura - come diciamo nella seconda mozione

È triste dover ammettere che le donne fanno notizia soprattutto se sono o vittime di violenza - e purtroppo sono tante le violenze, sempre di più - oppure veline. È così pervasivo il modello del velinismo, dell'esistere solo per la bellezza del corpo, che non posso non richiamare a titolo di esempio un episodio che riguarda un noto conduttore televisivo, Bruno Vespa, che mi ha molto colpita - si intende - negativamente. Presentando il Premio Campiello 2010, dove era arrivata finalista una giovane e brava scrittrice, Silvia Avallone, Vespa non trova di meglio che attirare l'attenzione del pubblico e delle telecamere sul suo *d**écolleté***. Morale: anche una scrittrice di talento viene trattata come una velina. del progetto europeo «Women and Media in Europe», ha dimostrato come l'immagine della donna offerta dalla televisione italiana sia stereotipata e molto spesso non corrispondente all'effettivo ruolo ricoperto dalle donne nella realtà della vita L'immagine prevalente è quella - si diceva in quel rapporto - patinata, sempre giovane e di bell'aspetto. Nei cinque anni che ci separano da quell'indagine le cose sono, se possibile, peggiorate, come ha documentato il video di Lorella Zanardo dal titolo

vedevano donne appese come prosciutti, immagini terribili oltre che offensive. Altro che rispetto della dignità! Allora, mi permetto di dire che quelle immagini sono sicuramente il frutto di una qualità scadente delle televisioni pubbliche e private, ma ciò succede anche perché la programmazione e i ruoli più importanti nelle televisioni sono nelle mani degli uomini. Lo sguardo in quei luoghi è tutto al maschile. primo dovere pubblico è migliorare la qualità della programmazione e dei palinsesti televisivi, adottando un severo codice di autoregolamentazione - come noi proponiamo nella nostra mozione - finalizzato al rispetto della dignità delle donne e alla valorizzazione della figura femminile in tutte le sue espressioni. Occorre poi riconoscere un maggiore peso di decisione alle donne e promuoverle nei ruoli più importanti. Nel nuovo Contratto nazionale di servizio si prevedono spazi nuovi e riconoscimenti per le donne; si prevedeva nelle nostre proposte, sostenute anche dalla senatrice Bonino, un osservatorio contro le discriminazioni e a tutela della dignità dell'immagine delle donne: peccato che questa nostra proposta

Il dispositivo impegna il Governo ad assumere il parere della Commissione di vigilanza in sede di stipula del Contratto di servizio tra Stato e RAI, quindi a svolgere un'opera di sensibilizzazione al rispetto della dignità delle donne; a rimuovere tutte quelle espressioni che indicano discriminazione nei confronti delle donne; a promuovere campagne finalizzate alla diffusione e alla valorizzazione del lavoro e delle opere delle donne in campo artistico, culturale, scientifico, politico; ad adottare campagne di sensibilizzazione nelle scuole, per aiutare i giovani a difendersi dai messaggi discriminatori nei confronti delle donne; a promuovere - questo è un impegno molto importante ma per noi molto più di valore - l'acquisizione di potere e di responsabilità da parte delle donne in tutti i settori della vita produttiva e sociale. È questa la premessa perché le donne vengano davvero rispettate nella loro dignità e nella loro

Signora Presidente, signora Ministro, il contesto generale è stato illustrato dalla collega Franco; interverranno altre colleghe, e oso persino sperare che intervenga qualche collega maschio. Fosse mai che vi interessi, fosse mai che vi sentiate in qualche modo coinvolti, anche perché il tema di cui discutiamo, che sia la rappresentazione al femminile nei *media* o nella pubblicità, ha appunto anche in conduttori maschili una serie di responsabili. Sono stata un po' incerta se presentare questa mozione, un po' perché la ritualità mi innervosisce e un po' perché ho sempre l'impressione e la paura - temo si verificherà anche questa volta - che, al di là del grande impegno o dei grandi discorsi, alla fine, anche quando si chiede una cosa

è una cosa, ripeto, apparentemente piccola, però significativa, sia sul piano istituzionale che su quello del merito.

che sia istituito un Osservatorio che, come in altri Paesi europei, monitori in modo terzo, professionale e indipendente la rappresentazione delle donne italiane nel servizio pubblico televisivo. È evidente, occorre un'analisi non di parte: io ho una posizione, un'impressione, una convinzione su come vengono rappresentate le donne italiane, però può darsi che ci servano dei dati più certi. Sono sicura che scopriremmo una ruolizzazione insopportabile; però, per fare una politica diversa, non proibizionista, non parruccona e neanche moralista, è importante avere un ente terzo, professionale e indipendente, che sia in grado di tracciare un panorama della situazione e anche di dare indicazioni su codici di condotta, su altri tipi di strumenti leggeri perché questa immagine venga modificata o, meglio,

lo dico per chi è della mia generazione, perché, personalmente, una *soap opera* di 350 puntate non mi condiziona più di tanto: lo dico perché i ragazzini e le ragazzine, di fronte a questo strumento, che peraltro è uno strumento

è come se le donne immigrate fossero tutte sostanzialmente delle poveracce. Non è vero: ormai abbiamo donne immigrate che sono *manager*, capi di imprese e di servizi. Insomma, tutto il mondo al femminile è schiacciato su due ruoli che assorbono quello che invece è molto più vario, molto più vivace e molto sottovalutato, anche perché a volte ci autosottovalutiamo. A volte siamo A volte siamo noi stesse che ci autosottovalutiamo e ci autocensuriamo, ed è come se i i tratti distintivi dell'essere femminile dovessero essere l'obbedienza, la pazienza e la disciplina, tant'è vero che l'aggettivo «ambizioso», che per un uomo è normale, appena si applica ad una donna diventa quasi un difetto.

obiettivamente ed evidentemente il marito se n'è andato, i figli le crescono storti; il marito che se ne è andato si è risposato con l'angelo del focolare, che ben che vada

appena pretendono qualcosa di più diventano veramente antipatiche e si capisce che, se le rappresentano così, giustappunto, il marito se n'è andato ed ha trovato la commessa. C'è quindi questo stereotipo per cui saremmo nate con un DNA un DNA che è più accogliente e più rumoroso; ma non è vero niente: è semplicemente che, come impariamo a stirare, impariamo ad occuparci, per dovere a volte, di tutto quello che gli uomini di questo Paese sono troppo occupati per seguire: avete troppo da fare

e siccome non è più così sarebbe bene che almeno il servizio pubblico riuscisse a dare ai nostri, e vostri, figli e figlie un'immagine un pochino più complessa della realtà italiana.

Ripeto: non voglio leggi proibizioniste, non voglio proibire proprio niente; non voglio vestire le persone e non le voglio manco denudare. Voglio semplicemente che siano rappresentate anche quelle che vanno in giro normalmente vestite, che hanno una professionalità, che sanno di merito, che sanno studiare, e così via. Cosa è successo? è successo? La Commissione di vigilanza, in modo assolutamente *bipartisan*, approva questo parere, che arriva al negoziato tra il Governo e la RAI;

niente trasparente, di cui non si capiscono i criteri, e che darà i risultati non apertamente, ma agli organi preposti, che non si sa manco quali siano.

che questo strumento di conoscenza, e questa fotografia, che sarà impietosa, forse faranno riflettere anche l'elemento maschile, preponderante, non solo al Senato, ma nelle posizioni di potere nel nostro Paese.

si può forse cercare di stimolare anche i pubblicitari, soprattutto il servizio pubblico, ad essere un po' più innovativi, anche un po' più tecnologici, anche un po' meno scontati.

femminile. Oggi la presenza delle donne sulla carta stampata e in televisione è più forte e più qualificata, oltre che numericamente più rilevante rispetto al passato; tuttavia non si può parlare ancora, neanche in questo, di una piena parità per le donne, che pure rivestono un ruolo strategico. È evidente che questa crescita non si può tramutare in motore di cambiamento fino a quando queste professioniste della comunicazione non si troveranno nelle condizioni di governare il processo decisionale, data la loro scarsa presenza in posti di rilievo. È la questione che abbiamo trattato anche oggi in Commissione finanze, che riguardava appunto di garanzia sulla presenza delle donne nei consigli di amministrazione, perché il tema è evidentemente sempre questo: la presenza femminile in luoghi decisionali. L'altra parte della mozione riguarda invece, come dicevo, la rappresentazione dell'immagine femminile. Di questo ci stiamo occupando da anni. Ricordo che anni fa, nel 2003 o nel 2004, era stata addirittura costituita una commissione, comunicazione e ruolo della donna, tra il Ministero della comunicazione ed il Ministero per le pari opportunità. Quindi è un tema che è fortemente presente. È di ieri anche il richiamo del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha affermato che è necessario incidere essenzialmente sulla cultura diffusa, sulla concezione del ruolo della donna, sugli squilibri persistenti e capillari nelle relazioni tra i generi, su un'immagine consumistica che la riduce da soggetto a oggetto, propiziando comportamenti aggressivi che arrivano fino al delitto. Questa è la situazione. È evidente che uno sguardo attento a come la figura femminile viene rappresentata nella pubblicità può dare indicazioni sul ruolo che viene assegnato alla donna in alcune circostanze, e in Italia la

style* è dura, ironica, vince premi a Cannes, senza però l'uso del corpo delle donne. È infatti la pubblicità banale, quella che non crea e non innova, che ha sempre bisogno di un uso del corpo femminile e sceglie quindi

utile a rimuovere le discriminazioni di genere tuttora esistenti nel campo della comunicazione e dell'informazione, proprio per rimuovere gli ostacoli che non permettono ancora alle donne, a tante brave giornaliste, a inviate di guerra, di arrivare ai luoghi decisionali e quindi di decidere cosa trasmettere o meno e come e quando e in che orari. Ciò dovrà essere fatto con campagne pubblicitarie di sensibilizzazione, attraverso il sistema radiotelevisivo e la carta stampata, che promuovano poi che promuovano poi il rispetto delle donne e della loro dignità. Proponiamo di predisporre una sorta di *vademecum* o di codice di autoregolamentazione che, nel rispetto della nostra cultura giuridica e costituzionale, elenchi le linee guida cui il servizio pubblico di informazione radiotelevisivo e della carta stampata dovrebbe uniformarsi per reintrodurre, anche nelle forme del linguaggio (lo sottolineo), il rispetto della persona di sesso femminile. Sarà evidentemente necessario coinvolgere le giovani generazioni, promuovendo anche nelle scuole campagne di sensibilizzazione proprio per diffondere un messaggio culturale di effettiva parità fin dalle scuole per valorizzare il ruolo delle bambine, delle ragazze e poi delle donne e rimuovere quegli stereotipi. Si chiede inoltre di intraprendere iniziative per individuare, riconoscere e premiare ogni progetto pubblico o privato che contribuisca a valorizzare la figura femminile ed il ruolo della donna nella società. Per questo, è fondamentale rafforzare ulteriormente il rispetto del principio di pari opportunità costituzionalmente sancito, intraprendendo tutte le azioni necessarie per valorizzare in ogni campo e ambito lavorativo la capacità ed il senso di responsabilità che il mondo femminile possiede e manifesta in tutti i settori, proprio per consentire una reale possibilità di

nelle mozioni che oggi stiamo presentando e discutendo, nel settore radiotelevisivo, in modo da favorire anche le donne nei ruoli apicali.

Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, il tradizionale conflitto tra vecchie e nuove generazioni oggi sembra essere diventato più stridente e aver assunto un ruolo centrale nella vita della nostra società. Si tratta di un fenomeno dovuto senza dubbio ai radicali mutamenti in atto, che ci sembrano aver investito soprattutto il rapporto tra famiglia, figli e istituzioni scolastiche, e che rischiano però ora di mettere a repentaglio modelli educativi consolidati e persino le fondamenta della nostra cultura. D'altra parte, quando si discute di trasformazioni della natura umana e della società, è inevitabile parlare di innovazione e rintracciare il fattore decisivo nell'avvento dell'era tecnologica. Ma sarebbe senz'altro più giusto e corretto interrogarsi sull'utilizzo di tale tecnologia. Così, nel corso degli anni, il cattivo uso della televisione ha creato uomini e donne, ma soprattutto giovani, forgiati da una civiltà dell'immagine che, lungi da essere uno strumento più immediato e diretto per comprendere il presente, pare essersi trasformata nella semplice ansia del vedere e del vedersi. Una modalità nella quale il sapere e il capire si riduce all'ambito delle cose visibili, a una rappresentazione fine a se stessa che ha impoverito non poco il mondo dell'astrazione e rischia di tradursi in idee prive di significato e di ancoraggio nel reale. In aggiunta a tale fenomeno, Internet, le comunità virtuali, i *social network*, e la sempre maggiore convergenza multimediale, hanno determinato una crescente pervasività nella vita delle persone, soprattutto dei giovani, e nel sistema delle relazioni interpersonali. Si è creata una generazione di ragazzi e persone non più abituate a relazionarsi dal vivo, a vivere nella comunità degli uomini e delle donne reali, quanto piuttosto abituate alla virtualità di una semplice connessione: omologata, fredda, priva di responsabilità sociale e per lo più basata sull'eccentricità fine a se stessa. Questi fenomeni sono in atto, ed è giusto sottoporli alla nostra attenzione per la pericolosità epocale che essi rivestono, ma ritengo utile che a questo punto ci si possa anche chiedere se la maggioranza del nostro Paese sia rispondente a questa rappresentazione, se insomma siamo davvero diventati così. Io penso di no, anzi, ritengo che la crescente incidenza di tali mutamenti - e la loro stessa pericolosità - abbia determinato il consolidarsi di una rappresentazione della società italiana che non corrisponde alla realtà, ben più complessa di come gli stessi giornali, la stessa televisione e lo stesso *web* tendano a rappresentarla. Il progresso della tecnica e della comunicazione è inevitabile, ma credo che esso vada sempre in qualche modo controllato e indirizzato - e vi prego di interpretare in maniera corretta questi termini - altrimenti potrebbe produrre effetti estremamente negativi. I modelli attuali - nei *media*, nella politica, nel mercato, nel costume - non mi sembra che stiano aiutando uno sviluppo positivo; piuttosto sembra stiano mettendo a dura prova, anche di recente, i principi su cui la nostra società si regge. In un contesto del genere, il perseguimento di una condizione di pari opportunità attraverso lo strumento illusorio della banalizzazione e relativizzazione dei costumi, retaggio del ha determinato la tendenza a un uso improprio della figura femminile e a una sua inappropriata rappresentazione da parte dei mezzi di comunicazione di massa (in proposito sono pienamente d'accordo con la presidente Bonino). Basti pensare alle pubblicità, con l'utilizzo del corpo femminile, maschile e persino infantile che sembra rivelare piuttosto l'incapacità del pubblicitario a trovare argomenti sostenibili e soluzioni creative in grado di impattare ed essere convincenti con gusto e originalità. È quindi una debolezza, una mancanza di fantasia, una povertà di idee che credo vada frenata e rigettata. Ecco perché oggi sembra più che mai necessario

come negli altri strumenti di comunicazione di massa, di immagini del corpo delle donne e degli uomini e di atteggiamenti e modelli a senso unico. Oggi più che mai ci sembra indispensabile uno speciale impegno nell'ambito dell'educazione. siamo di fronte ad un'emergenza educativa, è allora essenziale affrontarla con tutti gli strumenti che possiamo mettere in campo. Con questa mozione impegniamo quindi il Governo a promuovere ogni iniziativa utile a valorizzare il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa quali strumenti educativi e di formazione, evitando il rischio che la loro influenza possa porsi in termini concorrenziali o, addirittura, antagonisti, affinché, al contrario, si ponga in termini di integrazione e cooperazione con le agenzie educative tradizionali. inoltre, di adottare ogni iniziativa utile a promuovere, nell'ambito della comunicazione massmediatica, una rappresentazione della persona, della famiglia, delle agenzie di educazione e socializzazione il più possibile aderente alla realtà della società italiana e ai suoi principi fondanti. Infine, chiediamo di promuovere in ambito comunicativo la valorizzazione della figura femminile e una sua adeguata rappresentazione a tutto tondo che prescinda da modelli fittizi e da impropri stereotipi. La preghiamo, dunque, signora Ministro, di continuare nel suo ruolo e con le sue azioni fondamentali. Grazie Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha voluto approfittare di questo dibattito incentrato sul ruolo delle donne per affrontare una problematica specifica che permea la nostra società, ossia la presenza diffusa di stereotipi sessisti veicolati da messaggi pubblicitari che offendono e sviliscono le donne. Prima di continuare voglio, però, evidenziare che dispiace affrontare questo dibattito proprio nella settimana in cui ricorre la festa della donna, come se prima di oggi il problema non fosse stato altrettanto urgente.

Quello che innanzitutto chiediamo al Governo è di fornire una risposta concreta alla lotta contro le discriminazioni di genere perpetrate sotto forma di utilizzo di immagini che trasmettono, non solo esplicitamente ma anche in maniera allusiva, simbolica, messaggi che suggeriscono, incitano o non combattono il ricorso alla discriminazione, alla ridicolizzazione e all'offesa delle donne. Si finisce cosi per rappresentare il genere femminile - permettetemi di dirlo - come un esercito di prostitute e gli uomini come un esercito di utilizzatori finali. Una situazione non molto lusinghiera, in entrambi i casi. Oltre alle donne, dovrebbero sentirsi offesi da messaggi di questo tipo anche gli uomini. Eppure, sono poche le voci che si levano - purtroppo da entrambe le parti - per protestare. È evidente a tutti, ad esempio, che nonostante le segnalazioni dei consumatori, i richiami del giurì della pubblicità e le denunce di associazioni femminili attive sul campo, cartelloni stradali, giornali e televisioni ne sono ancora pieni con una frequenza e una ripetitività che fanno dell'Italia un caso di studio. L'immagine femminile viene utilizzata con elevata frequenza per pubblicizzare un ampio numero di prodotti che spazia dagli alimenti, ai prodotti di bellezza, alle automobili e via dicendo. Gli studi sulla rappresentazione dei generi nella pubblicità, ed in particolare sul ruolo della donna, hanno avuto un rapido sviluppo a partire dagli anni Settanta. Tali ricerche hanno evidenziato che, nell'ambito della pubblicità, in modo più marcato negli spot televisivi, è presente una forte discriminazione tra la rappresentazione degli uomini e delle donne. L'aspetto che emerge in modo più significativo è che, sebbene si cerchi di offrire l'immagine di una donna indipendente e sicura di sé, viene invece presentato il modello della donna oggetto, lasciando passare così, in modo più o meno velato, l'inferiorità del genere femminile rispetto a quello maschile. Esistono delle vere e proprie tecniche a forte contenuto psicologico che vengono utilizzate nell'elaborazione e nella costruzione dei messaggi pubblicitari. Si procede così alla frammentazione del corpo femminile; si mostrano solo alcune parti, rendendo il corpo un mero oggetto. Si assiste all'annullamento della donna in quanto persona si attua un processo attraverso cui la modella passa da soggetto ad oggetto, prendendo così il posto dell'oggetto che pubblicizza, che al contempo si umanizza. Crediamo sia giunto il momento di porre fine a questo fenomeno, che - lo ripeto - lede la dignità umana, senza distinzioni di genere. Chiediamo al Governo di mantenere ed onorare gli impegni già assunti dall'Italia nelle sedi internazionali e comunitarie. Gli interventi di organismi sopranazionali infatti non sono mancati in questo settore, ma purtroppo sono rimasti negli anni per lo più disattesi. Già nel 1997, con la risoluzione sulla discriminazione della donna nella pubblicità, il Parlamento europeo aveva constatato che la legislazione degli Stati membri in materia di protezione contro una rappresentazione degradante della donna nei mezzi di comunicazione era insufficiente; invocava un codice di condotta in questo settore. La risoluzione del 1997 sottolineava che lo sfruttamento ingiustificato del corpo femminile a fini commerciali può offendere in modo particolarmente grave la dignità della donna, e ribadiva quanto i mezzi di comunicazione di massa siano in grado di influenzare i comportamenti sociali attraverso i modelli trasmessi, nonché contribuire a un cambiamento della mentalità e alla realizzazione dell'eguaglianza rappresentando la varietà di ruoli dei due sessi. Ancora nel 2008, sempre il Parlamento europeo si è espresso nuovamente sull'argomento ha emanato una proposta di risoluzione sull'impatto del *marketing* e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini. Con tale atto si invitava il settore della pubblicità a rinunciare interamente a sminuire la donna a oggetto sessuale; si chiedeva altresì agli Stati membri di incoraggiare il settore pubblicitario a dar prova di maggiore e più costruttiva creatività nell'ideazione della pubblicità, per evidenziare l'importanza della donna per la società nel lavoro, nella famiglia e nella vita pubblica. Facendo un passo indietro, nel 2005 il Comitato ONU per l'attuazione della CEDAW (Convenzione per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne) raccomandava di adottare un programma su larga scala, onnicomprensivo e coordinato, per combattere la diffusa accettazione di ruoli stereotipati di uomini e donne. nessun atto concreto e realmente efficace è stato adottato a riguardo, nonostante l'importanza accordata da tutti i Governi al problema. Affrontare il tema della distorsione degli stereotipi femminili nel mondo della comunicazione è un'occasione importante per crescere ed evolvere. Attualmente, la materia viene autoregolata dagli operatori del settore pubblicitario tramite l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP), il cui codice della comunicazione commerciale è vincolante per i soggetti che operano nel settore delle comunicazioni e che lo hanno sottoscritto. Nel codice di autodisciplina si dice chiaramente che i messaggi devono rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e devono evitare ogni forma di discriminazione. A seguito di questo principio, sono state vietate alcune pubblicità particolarmente offensive, che evito di citare perché troppo indegne. Il problema è che la nostra legislazione è più blanda di quella di altri Paesi europei soprattutto, c'è una minore sensibilità delle parti in causa, soprattutto dei committenti e dei pubblicitari. Lo IAP rappresenta diverse sigle del mondo pubblicitario, ma non può essere l'organo deputato al monitoraggio della comunicazione pubblicitaria nella sua interezza. C'è bisogno di un intervento normativo

Solo così si potrà giungere ad un'informazione pubblicitaria rispettosa della figura femminile, provvedendo a colmare una grave lacuna del nostro ordinamento legislativo. Porre un freno alla pubblicità sessista è doveroso nei confronti della stragrande maggioranza delle italiane, studentesse, lavoratrici e casalinghe, soprattutto oggi che, a seguito degli eventi degli ultimi mesi che hanno coinvolto una sparuta minoranza di donne che si è offerta come merce, e come tale è stata considerata, c'è il rischio che si rafforzino nell'immaginario collettivo pregiudizi e stereotipi. Concludendo, signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei invitarvi invitarvi a non sottovalutare l'occasione di riflettere sul ruolo che le donne rivestono oggi in Europa, nonostante le molte difficoltà, e al contempo sulla situazione delle donne italiane, di certo non rosea, come ha avuto modo di dirci ieri il presidente Napolitano. Per questo chiediamo al Governo un impegno concreto per recepire il prima possibile le indicazioni europee e internazionali; per istituire un organismo pubblico volto al contrasto della discriminazione della donna nei *media* e nella pubblicità; per promuovere, attraverso il sistema radiotelevisivo pubblico, la diffusione di un'immagine diversa della donna, in particolare per quel che riguarda il suo inserimento nel mondo del lavoro. Infatti, il mercato del lavoro rischia di subire una fortissima inversione di tendenza a netto svantaggio delle donne, che negli ultimi anni avevano cercato di lottare contro la disoccupazione e l'inattività. La crisi economica non ha fatto altro che peggiorare la situazione delle lavoratrici. Il numero delle donne occupate è fermo al 46 per cento circa contro il 60 per cento che si sarebbe dovuto raggiungere ben due anni fa, secondo gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea a Lisbona, mentre l'occupazione degli uomini è pari al 68 per cento. Di tutto questo non si parla, o si parla molto poco, sui *media*. Sarebbe interessante promuovere una campagna che ricordi che il tasso di occupazione delle donne è nettamente inferiore rispetto a quello degli uomini; che il grado di incidenza che la precarietà del lavoro ha sulla vita delle donne è pari al doppio di quello degli uomini; che il persistere della differenza salariale continua a far sì che le retribuzioni delle lavoratrici donne, a parità di mansioni, siano inferiori a quelle dei colleghi uomini. apre una nuova finestra"). Colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti della Scuola statale «Montessori» di Roma, ai quali diamo il benvenuto.

L'Europa sta infatti attraversando un periodo difficile dovuto alla crisi economica e finanziaria. Tale crisi, a nostro avviso, può e deve essere contrastata anche attraverso il potenziamento di un sistema di garanzie che fondi le sue radici sulla valorizzazione di quei principi che hanno rappresentato il valore aggiunto che ha consentito la costruzione di un Paese civile in grado di essere motore di benessere e di crescita di una società sana. valori quali la famiglia - quella tradizionale - il senso di appartenenza alla comunità, al territorio in cui si vive, l'essere consapevoli che ogni cittadino deve restituire alla comunità alla quale appartiene azioni che favoriscano il bene comune. Non dimentichiamoci i valori che afferiscono al rispetto ed alla dignità delle persone. purtroppo vivendo in un'epoca dove trionfa il relativismo, l'individualismo, dove l'etica non è più un bene che nutre la comunità, ma è diventata una pratica facoltativa. La globalizzazione sta erodendo l'identità, le radici storiche e culturali, le tradizioni, il senso di unione e di solidarietà tra le persone, e soprattutto il valore etico del rispetto per la persona, per le donne in modo particolare. Tutto ciò si può riscontrare in modo particolare ed evidente nell'ambito della comunicazione multimediale: certamente in grado di offrire una molteplicità di informazioni e saperi a disposizione di tutti, ma anche, contestualmente, per la possibilità di incidere fortemente sulla formazione della società odierna divenendo strumento di liberazione di saperi e conoscenze ed insieme strumento di controllo sociale in modo semplice, veloce ed esteso. la comunicazione multimediale non può che rispecchiare e moltiplicare il relativismo, l'individualismo, la concezione che l'etica non è più un bene collettivo che aiuta a crescere, ma un *optional* da usare se e come conviene e, quindi, la possibilità che tutto, ma soprattutto la dignità delle persone e delle donne in particolare, possa essere mercificata, essere oggetto di violenza e piegarsi all'interesse personale del momento, perdendo di vista - lo ripeto - il bene comune. È chiara la responsabilità di buona parte della comunicazione multimediale, (pubblicità, spettacoli di intrattenimento, cinematografia e quant'altro), nel determinare proprio la tendenza ad uso strumentale della figura femminile, ad una sua rappresentazione tesa a negare quella dignità di cui ha diritto, quel riconoscimento delle caratteristiche che la distinguono e la innalzano. È altrettanto chiaro che buona parte di quella comunicazione multimediale negativa è di fatto richiesta da un vasto pubblico che, impreparato alla capacità di riflessione critica nei confronti di questa realtà, se ne abbevera e la subisce più o meno inconsapevolmente.

Siamo in presenza di un circolo vizioso che si autoalimenta, di un gatto che si morde la coda, incapace di fermarsi e di riflettere. Per questo motivo, la Lega Nord chiede al Governo di promuovere ogni iniziativa utile anche a valorizzare e potenziare gli strumenti di educazione dei giovani ad un utilizzo critico, consapevole e responsabile della comunicazione multimediale. È emerso anche da un'indagine Grazie che gran parte delle famiglie dei nostri studenti non utilizza, o utilizza rudimentalmente, Internet e la comunicazione multimediale, e che i nostri giovani usano molto bene e velocemente questi strumenti, ma non conoscono il codice dei linguaggi degli stessi e, quindi, non possono porsi con senso critico rispetto ad essi. La Lega Nord chiede al Governo anche di adottare ogni iniziativa utile ed adeguata affinché la comunicazione multimediale rappresenti la persona, la donna e la famiglia per quello che sono nella realtà quotidiana, in modo tale che i valori di una società sana ritornino in primo piano e, in modo particolare, che alla donna venga riaffiancato il valore aggiunto di cui essa è portatrice nella nella comunità. Tutto ciò per la Lega Nord può rompere l'autoalimentazione del circolo vizioso di cui ho parlato prima, può fermare quel gatto che si morde la coda.

Ministro, cerchiamo di fare quadrato oggi sui contenuti in discussione. È una grande occasione per dare un messaggio molto chiaro e preciso al Paese, a quelle donne e a quegli uomini indignati, ma anche a coloro che sono confusi.

questo strumento di informazione rappresenta di fatto la fonte principale di formazione, individuale, di massa e quindi collettiva.

una grande occasione di esercitare una delle sue funzioni fondamentali: quella di porre al centro dell'interesse di chi ha responsabilità di governo - quindi mi rivolgo a lei, Ministro e quindi di indirizzo delle pubbliche istituzioni, questioni che mostrano elementi degenerativi del modello di società su cui si fonda il vivere civile. Oggi, ciò è reso ancora più urgente dalla distanza che viene percepita dai cittadini tra la politica e i problemi reali della vita quotidiana. Tale dicotomia raggiunge la sua massima espressione proprio sui temi contenuti nelle mozioni: una dicotomia che nasce dalla tradizionale rappresentazione virtuale distorta che i mezzi di comunicazione offrono della donna rispetto al ruolo insostituibile che essa svolge nella società. L'immagine della donna, come ha detto ieri il presidente Napolitano, più oggetto che soggetto, che fa della bellezza e della giovinezza i parametri del proprio successo, non è l'icona di una rappresentazione teatrale che lo spettatore osserva sapendo che essa si esaurisce con la conclusione dello spettacolo. Nella vita reale, le donne vere sono quelle che prestano cura, lavorano, studiano, si impegnano per garantirsi una carriera, spesso in condizioni di maggior difficoltà, per le quali l'affermazione della personalità avviene con percorsi di sacrificio e non sempre giunge a completamento per i troppi ostacoli nel lavoro, nella famiglia e nella società. Ma quell'immagine virtuale è uscita della scatola; quelle donne sono diventate reali nel momento in cui nella coscienza delle persone diventano modello. Tale confusione - e uso un termine delicato - ha introdotto nel nostro Paese una cultura che è la risposta mancata alle prospettive di futuro delle ragazze e dei ragazzi italiani. L'impossibilità di costruire un progetto di prospettiva fondato su studio, lavoro ed opportunità di vita autonoma ha lasciato ampio spazio alla rappresentazione mediatica ed illusoria della via breve per il successo, del denaro facile, che diventa il lasciapassare anche nelle professioni. I modelli virtuali si sono mescolati con quelli reali e le aspirazioni, i comportamenti, i rapporti tra uomini e donne ne sono sempre più condizionati: le malattie del comportamento diffuse in molti bambini e bambine, le patologie alimentari, l'aumento della violenza sulle donne, estesa a tutti gli strati della società, sono campanelli d'allarme che suonano da tempo. Sicuramente, le cause non sono da ricercarsi solo in quest'ambito, ma è sicuramente nel rapporto tra *media* e coscienza individuale che hanno trovato la più ampia cassa di risonanza, ed è qui che bisogna porvi rimedio provocando un'inversione del circuito. Meno virtualità nella realtà e più realtà nei *media*. Ma non solo cronaca: abbiamo bisogno che vengano trasmessi esempi positivi di donne che in carne ed ossa mostrino il proprio talento, modelli educativi che reindirizzino le legittime aspirazioni alla ricerca di un'autonomia attraverso le reali possibilità e non le effimere illusioni della strada facile. Credo che tale preoccupazione sia trasversalmente presente in tutte le mozioni e in tutte le le madri, e i padri, che, faticosamente, ogni giorno, lottano per l'educazione dei propri figli e delle proprie figlie contro un'idea distruttiva opposta al loro insegnamento; coloro che non sono in possesso degli strumenti critici necessari, la questione è ancora più complicata e difficile, perché li confina in una trappola senza uscita. È dunque fondamentale nelle responsabilità di chi governa ottimizzare l'uso degli strumenti a disposizione. Nel dispositivo contenuto nella nostra mozione vengono indicati impegni possibili e precisi, che possono realmente incidere sulla diffusione di un nuovo, e anche ritrovato, rispetto della dignità della donna nella sua diversità, perché solo da qui può trovare spinta l'avvio di un nuovo umanesimo, che riporti al centro la persona in sé. Da qui potrà poi ripartire quel Rinascimento, che noi continuiamo tutti a chiamare cambiamento, tanto invocato e immaginato dal nostro Paese.

i problemi e le cose ancora da fare rispetto a una politica di parità e, al contempo, di valorizzazione delle differenze - perché questi sono i

Grazie

e su questo vorremmo che si impegnasse l'Assemblea. Assumere un punto di vista vuol dire guardare a questo universo femminile nella sua realtà, esaltandone le capacità, le competenze e il sistema valoriale che mette in campo per raggiungere gli obiettivi, a partire dai più modesti, che poi modesti non sono mai, nella consapevolezza -

Il tema che oggi mettiamo a fuoco ha due punti di riferimento, che credo vadano ricordati. Il primo, già evidenziato da altri in Aula, è la risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008

una straordinaria assemblea di donne nell'Aula magna dell'Università statale di Milano, organizzata dal Dipartimento di diritto della costituzionalista, che tutti conosciamo, Marilisa D'Amico.

che detto Osservatorio langue perché il contratto di servizio RAI non è stato firmato. Ministro, capisco che non è il suo settore

romane. Gli altri due elementi che hanno mosso nell'opinione pubblica una consapevolezza forte, ancora prima

con delle riviste italiane, le più qualificate riviste politiche italiane, ogni tanto vedono i colleghi stranieri che guardano e magari chiedono: vai in giro con un giornaletto un po' *cochon*? Non

che fa loro comodo non saperlo - di avere in mano uno strumento che veicola messaggi, valori, e che è più potente, purtroppo,

figli dei valori che abbiano la forza di resistere alla potenza che viene da questi mezzi, che essi usano in maniera unidirezionale. Forse la salvezza sarà

In conclusione, noi chiediamo di firmare il contratto di servizio RAI, nel quale c'è l'Osservatorio, e quindi che tutte le persone che credono alle cose che diciamo se ne facciano promotrici; di fare campagne di questo genere;

di trasmettere con tutte le campagne possibili il punto di vista che deplora socialmente chi si comporta in un certo modo. Nei Paesi dove funzionano queste cose ciò avviene perché c'è un livello di coscienza e di consapevolezza tale per cui c'è la deplorazione sociale, nel senso che chi si comporta così si comporta male.

e di conseguenza anche a quelle politiche. Quello che finora non abbiamo avuto il coraggio di dire con grande franchezza in questo ricco dibattito, dove spero di sentire anche qualche voce maschile partecipare al confronto

e che là dobbiamo cercare innanzitutto le risposte alle dolorose domande che anche la senatrice Adamo si è posta nel suo ultimo intervento, perché là troviamo le possibili soluzioni. Cosa voglio dire esattamente? Voglio dire che quello che è entrato in crisi attraverso l'immagine della della donna nei vari sistemi della comunicazione, innanzitutto della pubblicità così come molto altro - e di molto altro vorrei parlare - è il nostro stare al mondo, nel mondo, e il nostro essere oggi cittadini e cittadine, in uno schema dove quotidianamente arretriamo dal ruolo di cittadini e cittadine ed entriamo sempre di più, e sempre più a pieno titolo, nel ruolo di consumatori e consumatrici. Penso

quanto invece assecondiamo il nostro stare nella società da consumatori. Questo cambia completamente la prospettiva, perché fino a quando riusciamo a tenere forte il ruolo del cittadino rispetto a qualsiasi altro ruolo, giustifichiamo e continuiamo a dare valore e significato persino a quest'Aula e cioè alla rappresentanza di quel cittadino e di quella cittadina. Invece, abdicando quotidianamente a questo, spostiamo la rappresentanza di quelli che diventano sempre meno cittadini e sempre più consumatori; e la rappresentanza a quel punto spetta alle associazioni dei consumatori e non più alla rappresentanza civica e politica, della quale noi qui siamo l'espressione. È allora la persona e la sua declinazione di cittadino e di cittadina che ci devono interessare, ed è la coesione sociale (alla quale dovremmo tutti aspirare, lavorando qua dentro per costruirla e cementarla) che ci chiama all'obbligo di ricondurre sul fronte della rappresentanza civile il tema della coesione sociale.

continuare a trattare a fasi alterne e a corrente alternata, per cui il giorno che ci torna comodo è frontiera di libertà e il giorno che ci torna meno comodo è invece il luogo oscuro dove l'immagine negativa che non vorremmo mai vedere, come quella che la senatrice Adamo ha ha citato così bene e che campeggia nell'atrio della stazione di Milano, produce i suoi effetti sulle persone più deboli della nostra società, sulle famiglie meno attrezzate, su tutti coloro che dovremmo difendere e aiutare ad elevare la propria condizione di cittadino e di persona dentro una comunità e quindi una società. società. Ha ragione la senatrice Adamo quando dice che è una battaglia contro gli stereotipi, tutti gli stereotipi, non solo questo; non è la nota marca di slip che si propaganda alla stazione di Milano l'unico stereotipo, ce ne sono tanti tutti concorrono a questa visione consumista della nostra vita. Pochissime di queste immagini aiutano ad ancorarsi ad un sistema di valori dove la persona (la persona-bambino, la persona-donna, la persona-uomo) vive la propria condizione da protagonista di una comunità e di una società.

dove spesso continuiamo a far rotolare alcune immagini di generazione in generazione. Oggi siamo di fronte alla forza e alla potenza dei sistemi di comunicazione. Guardo con grande attenzione, e anche con qualche sospetto, ai messaggi, assolutamente fuori controllo - perché quella non è più libertà, è essere oltre la libertà - di Internet, che mi preoccupano forse più ancora di quelli televisivi, perché lì è ancora più pervasiva e oscura non solo la trasmissione, ma la formazione di quella immagine, di quel pensiero, di quella comunicazione, poiché non controllata da nessuna parte e soprattutto originata da pensieri che non sempre possono subire il vaglio della trasmissione corretta della comunicazione, dei valori, degli insegnamenti di ciò che viene trasmesso e comunicato. Allora, riguardo alla comunicazione farei uno sforzo in quest'Aula del Parlamento, chiedendo alla nostra Commissione di vigilanza sulla RAI di cominciare ad occuparsi non solo dell'immagine femminile o degli stereotipi sbagliati che spesso la televisione di Stato manda in onda, ma di tutti i messaggi Noi dobbiamo oggi interrogarci se ci basta occuparci della scatola nera che sta nelle nostre case, o se invece dobbiamo cominciare ad occuparci anche di quella scatolina più piccola che sta nelle tasche di tutti i nostri giovani e fare in modo che la Commissione di vigilanza possa vedere estesi i suoi poteri anche a quella forma di comunicazione, perché questa può essere la risposta moderna ad una rapidità che ci sta travolgendo tutti, mentre noi siamo ancora fermi alla televisione di qualche decennio fa ed alla Vigilanza di qualche decennio fa. Vorrei complimentarmi col ministro Carfagna, che ieri, dal Presidente della Repubblica, in occasione della celebrazione internazionale della donna, quella che ricordiamo ogni 8 marzo, ha saputo portare non solo l'elenco, numeroso, delle tante iniziative positive che questo Governo ha potuto dedicare alle donne italiane, ma anche ricordarci una lunga lista di cose buone, fatte da donne prima di noi in quest'Aula o nell'altro ramo del Parlamento a favore delle donne italiane. vorrei complimentarmi col ministro Carfagna per tutto il lavoro svolto, insieme alla maggioranza innanzitutto, ma molte volte anche con molte parti dell'opposizione, riesce a realizzare a difesa delle donne italiane, traducendo quelle azioni positive dalle quali tutte partiamo e vorremmo vedere messe in campo in atti forti, importanti, di leggi che piano piano stanno cambiando la vita delle italiane. È inutile che ricordi io - sono certo che potrà farlo lei meglio di me - come la legge italiana sullo *stalking* sia una legge che oggi viene presa a modello da molti altri Paesi europei. Così come vorrei poter dare, non solo alla senatrice Adamo ma a tutta l'Assemblea, la comunicazione formale, nell'ufficialità dell'Aula, che solo un'ora e mezza fa la Commissione finanze ha concluso il suo lavoro

atto possibile, non solo in occasione di questo 8 marzo e di questa settimana, ma nell'occasione quotidiana del nostro lavoro, nella traduzione di quelle azioni positive che hanno origine da lontano, il frutto delle lotte di tante donne prima di noi, che nella legge n. 125 del 1991 abbiamo per la prima volta celebrato negli atti normativi del nostro Paese, fino poi a tradurlo nella legge n. 215 del 1992 sull'imprenditoria femminile, e oggi, finalmente, in questa innovativa e potente legge che aiuta le donne a sfondare quel soffitto di cristallo che sta sempre sopra la loro testa nei consigli di amministrazione delle società, nella vita economica come nella vita sociale, a tradurre da azioni positive a leggi quello che è lo straordinario sguardo delle donne sul mondo che noi oggi, spero degnamente, siamo qui a rappresentare.

Signora Presidente, spero che l'invocato intervento di persone di sesso maschile non comporti necessariamente un aumento del brusio dell'Aula. Ho avuto

Ebbene, io, che non ho ragioni di avversità, né verso la bellezza, né verso la giovinezza, vi assicuro che quei 22 minuti di immagini pubblicitarie trasmesse dalla televisione italiana pubblica e privata sono definibili in un solo modo: devastanti. colleghe, i colleghi e la Presidenza del Senato a guardarlo, perché ci offre uno spaccato che, se fosse quello di tutta l'Europa, di tutte le televisioni del mondo civile, occidentale e non, forse sarebbe un po' più sopportabile. Ma non è così, colleghi, signora Presidente, perché i pubblicitari, gli inserzionisti e i creativi di altri Paesi che, al pari del nostro sistema televisivo, hanno nella risorsa pubblicitaria un aspetto fondamentale per la vita delle aziende e per la stessa libertà, non usano

è del tutto evidente che, se altrove è possibile costruire messaggi pubblicitari efficaci dal punto di vista del *marketing* e del pubblico a cui si rivolgono

meno belli dei nostri, non meno efficaci e accattivanti, ma anzi lo siano altrettanto se non di più, senza l'uso della volgarità e senza l'offesa alla dignità

a colpi di norme che si affastellano: è un problema gigantesco di natura culturale e politica, e dobbiamo sapere come affrontarlo.

di farsi promotore di incontri con gli operatori, con le aziende editoriali televisive pubbliche e private,

mentre sappiamo che anche nella realtà dei *media* sono sempre di più le donne protagoniste, anche in ruoli tutt'altro che trascurabili. Non è vero Non è vero che la donna nel nostro Paese sia solo un corpo da rappresentare nella pubblicità o una protagonista di episodi di cronaca nera. Non è vero: c'è anche questo, ma ci sono anche tante donne che hanno saputo affermarsi per ragioni meramente legate al talento, alle capacità e alla serietà del proprio lavoro. Cominciamo da qui. Concludo, signora Presidente, con un invito al Governo. Come è noto, la competenza nel nostro ordinamento per rivolgere indirizzi all'azienda di servizio pubblico. Tale competenza è del Parlamento, attraverso il lavoro della Commissione parlamentare di vigilanza; stipula il contratto di servizio a nome dello Stato. Lo Stato stipula il contratto di servizio con la RAI, che è tuttora in discussione,

il compito di fornire un parere che per il Governo è obbligatorio acquisire, anche se non è vincolante. In tale parere la Commissione, con il voto di tutti i commissari (di destra, di sinistra e ha accolto molte delle istanze che le colleghe donne dei due rami del Parlamento hanno avanzato. Ora, è importante che, anche in considerazione alle resistenze

"aperturista" della Commissione parlamentare di vigilanza, che non sappiamo ancora se diventerà testo nel negoziato tra il Governo e la RAI. C'è stato un rallentamento di mesi, e la firma non c'è ancora. Non c'è ancora il nuovo contratto di servizio, che contiene, magari ancora in modo insufficiente, misure certe a difesa della dignità della donna e per la promozione di un monitoraggio su come la televisione tratta questa

Senatore Morri, nel rispetto delle competenze delle istituzioni proprio da lei richiamate, la Presidenza del Senato si farà carico delle sue osservazioni. Presidente, le mozioni che discutiamo oggi sull'immagine della donna nei mezzi d'informazione

bisogna però evitare, su argomenti di questo genere, di scadere nel luogo comune, in omaggio all'argomento del giorno (anche se oggi non è più l'8 marzo). Il fatto Il fatto che vengano proposti con una certa insistenza modelli, stereotipi subalterni della donna che basano unicamente la personalità e le aspirazioni sull'aspetto fisico è sicuramente reale,

ne viene fatto), in generale, quali sono i giovani che ricevono attenzione dai mezzi di informazione? Se un giovane, maschio o femmina che sia, non è né calciatore,

per sostenersi agli studi (perché non tutti nascono con la possibilità di mantenersi) sono totalmente ignorati. Se invece si lamentassero, compissero un delitto, se partecipassero a qualche *reality show* dove

Un altro luogo comune che credo dovremmo evitare in quanto rappresentanti del popolo della Repubblica italiana è di scadere nel solito stereotipo del «solo in Italia

non possiamo certo paragonarli a certe trasmissioni leggere, e anche, nella pretesa, meno leggere della nostra televisione. Ma non esistono solo questi canali intellettuali di approfondimento;

che peraltro, da quello che risulta, non è è obbligato, ma è compensato adeguatamente, sia lesivo di tutti coloro che appartengono allo stesso genere.

ha certi comportamenti fuori dalle righe piuttosto che in una donna che ha altri comportamenti fuori dalle righe, poiché in entrambi i casi essi seguono degli stereotipi rigidamente maschili o femminili, ma solo perché devono interpretare la loro parte in commedia. Ebbene, io non sento la non sento la mia personale dignità lesa da questa persona perché appartiene al mio stesso genere, piuttosto che alla mia stessa categoria sociale, alla mia regione o ad altre

Parliamo ad esempio dei dibattiti politici, o presuntamente tali. Sappiamo bene che è molto più facile, e molto più diffuso, il dibattito a forza di urla, di *slogan* o

che il dibattito politico è fatto di approfondimenti molto più seri: c'è un atteggiamento, in generale, assai meno fatto di urla e assai più di collaborazioni, nell'ambito delle quali ci sono le contrapposizioni, com'è giusto e sano che sia per una democrazia rappresentativa. Eppure, esiste una rappresentazione falsata del mondo della politica, dove sembra che la giornata del politico, fatti salvi alcuni aspetti parapolitici, che non hanno nulla a che fare con la politica

reali che si affrontano si otterrebbe un'attenzione maggiore. Questo però è più costoso e richiede una maggiore fatica da parte delle redazioni, da parte di coloro che

nel parlare del tema donne e sistema dei *media* è importante a mio avviso ricordare a tutti noi che la dimensione europea delle politiche di pari opportunità ha registrato nel 2010 una vera svolta costituzionale nell'Unione europea. Infatti, l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha costituzionalizzato nel suo articolato i principi di uguaglianza, di parità, anche con azioni positive, di non discriminazione, di lotta a ogni forma di violenza, sfruttamento e tratta. Vorrei aggiungere che con la Carta delle donne l'Europa inserisce il diritto alla dignità, integrità e fine della violenza basata sul genere nel *corpus* normativo europeo. Questi nuovi diritti s'inseriscono in un'ulteriore evoluzione istituzionale che dà più poteri di colegislatore al Parlamento europeo e inserisce il cosiddetto terzo pilastro, lo spazio giuridico europeo della giustizia, sicurezza e lotta alla criminalità, all'interno dell'ordinamento europeo. Un ulteriore passo avanti è stato compiuto anche con l'approvazione da parte della Commissione europea della nuova «Tabella di marcia per la parità 2010-2015», mentre noi siamo ancora molto, molto lontani Un ulteriore passo avanti è stato compiuto anche con l'approvazione da parte della Commissione europea della nuova «Tabella di marcia per la parità 2010-2015», mentre noi siamo ancora molto, molto lontani dall'aver raggiunto gli obiettivi fissati nella precedente tabella. Inoltre, il Parlamento europeo ha approvato il 15 dicembre 2010 una risoluzione sull'impatto della pubblicità sul comportamento dei consumatori. La risoluzione evidenzia che lo sviluppo delle nuove pratiche pubblicitarie *on line* e via cellulare sta generando una gamma di problemi che devono essere affrontati per salvaguardare un alto livello di protezione degli utilizzatori. Sulla base del parere della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, nella risoluzione viene affrontata la tematica della parità di genere e della dignità umana nella pubblicità. La Relazione invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare provvedimenti adeguati per assicurare che la commercializzazione e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione basata sul genere, sulle convinzioni religiose, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. La pubblicità è uno strumento efficace per contrastare ed eliminare gli stereotipi, nonché un mezzo per combattere il razzismo, il sessismo e la discriminazione. In questa ottica, viene rivolto agli Stati membri ed ai professionisti della pubblicità l'invito a rafforzare le attività di formazione ed istruzione per superare gli stereotipi, a combattere la discriminazione ed a promuovere l'uguaglianza di genere sin dalla tenera età. la pubblicità divulga messaggi discriminatori e indegni, basati su ogni forma di stereotipo di genere, che ostacolano le strategie a favore dell'uguaglianza di genere. Per questo la Commissione invita gli Stati membri, la società civile e gli organismi di autoregolamentazione nel settore della pubblicità a collaborare per contrastare tali pratiche. La pubblicità dei beni di consumo è legata direttamente alla stampa, alla radio e alla televisione, di cui costituisce un elemento inscindibile, e indirettamente all'industria cinematografica e alle produzioni televisive sotto forma di commercializzazione dei prodotti; ciò consegue che una pubblicità affidabile e la promozione di sani modelli di comportamento possono avere un'influenza positiva sulla percezione, da parte della società, di tematiche quali ruoli di genere, immagine del corpo umano e normalità. Il Parlamento deve allora incoraggiare i pubblicitari a formulare messaggi più costruttivi, al fine di promuovere il ruolo positivo delle donne e degli uomini nella società, nel mondo del lavoro, in famiglia e nella vita pubblica. Ecco, cari colleghi, signora Ministro, un concreto quadro di riferimento da cui partire per dare un segnale positivo alle donne italiane, promuovendo l'acquisizione di *empowerment* e e l'istituzione di organismi deputati al monitoraggio e al controllo di quanto disposto dal Parlamento. Care colleghe, cari colleghi, il ritorno in campo delle donne in questi giorni afferma la necessità di una parità sostanziale ed esprime perciò una richiesta di azioni strutturali, una domanda di politiche attive e trasversali, perché soprattutto nell'era della globalizzazione, caratterizzata dalle molteplici appartenenze, questa è la priorità. Bisogna perciò smettere di considerare il tema delle donne di serie B e raccogliere piuttosto la sfida europea che offre una nozione di cittadinanza come quadro di garanzie, che estende la possibilità di libertà degli individui di muoversi tra molteplici opzioni e identità. È questa, vedete, vede signora Ministro, una straordinaria scelta per il cambiamento, che certo non potrà avvenire senza un ritorno in campo forte ed un'azione vigile e costante delle donne. Devono saperlo fare riconoscendo un superiore e comune interesse per ragionare senza alzare steccati, come voi state facendo. In definitiva, cara ministro Carfagna, penso stia proprio in questo l'importanza e il valore di quel grande movimento che si è realizzato il 13 febbraio scorso. In quelle piazze non c'erano né faziosità, né strumentalizzazione politica; c'era invece la necessità di un'Italia diversa, un'Italia di donne e di uomini con una forte identità nazionale, protagonisti nel processo di integrazione europea e al servizio di nuove relazioni tra popoli e Stati. Per questo, sui temi oggi alla nostra attenzione e su altri ancora sfidiamo e sfideremo il Governo nel merito, per garantire quel significativo passo avanti verso la tutela della dignità e la garanzia della parità uomo-donna, ancora ieri sostenuta con forza e autorevolezza dal Presidente della Repubblica.

La chiamerò così, anche se il suo nome era un altro, più nuovo e moderno. Maria era giovane, bella e di famiglia facoltosa. Viveva nella mia città: Napoli. Era frastornata da una certa sua fragilità e dalle migliaia di immagini che le rimbalzavano davanti agli occhi: donne patinate, bellissime, ammiratissime. Soprattutto, magrissime! Una di quelle immagini ha campeggiato sul suo frigorifero e l'ha tormentata per due anni. Il tempo che le è stato necessario per privarsi del dono più prezioso: la vita. Senza accorgersene, digiunando. Per assomigliare a quell'immagine da sogno.

E non è solo un modo per celebrare l'8 marzo. Il mondo femminile viene raccontato dai mezzi di comunicazione di massa, soprattutto dalle televisioni, in modo da fornire all'immaginario collettivo, in particolare ai giovanissimi ed alle giovanissime, uno stereotipo ingannevole, per molti versi dequalificante. E pericoloso. Ai tempi delle battaglie femminili e femministe si parlava di «esaltazione della donna oggetto», desiderato oggetto di sfruttamento sessuale o commerciale. Quante sono le pubblicità che, pure per propagandare prodotti che nulla - lo diceva prima la senatrice Adamo - ma proprio nulla hanno a che vedere con il corpo delle donne utilizzano immagini di donne nude, o in abiti succinti, o in pose provocanti e allusive? Tutto ciò non solo è pericoloso, perché detta modelli di comportamento distorti e che danno una visione altrettanto distorta della femminilità, ma è insopportabile, perché nasconde, ignora la vera realtà della vita delle donne, la loro vivacità, la loro professionalità, il loro essere madri e mogli, la dura fatica che tante volte mettono per tenere insieme i tanti ruoli che svolgono.

I *mass media* difficilmente raccontano le vite normali, difficilmente inquadrano i volti normali delle donne. Non si parla mai dell'impegno delle donne, dell'azione dell'azione delle donne, delle anziane, delle disabili, delle povere, delle disperate; a meno che non siano protagoniste di atti di violenza o di brutalità: ed allora, via ai dettagli macabri, ai *talk show*, ai plastici. Il nostro Paese ha diritto a un profondo cambiamento, a una televisione che parli delle donne normali, valorizzi ed esalti le competenze, i talenti e non solo il corpo delle donne, che educhi ad accettare la complessità,

stereotipi. Occorre contribuire ad avviare un'evoluzione culturale per una più realistica percezione del femminile. Credo che questo lo esigiamo tutte: lo dobbiamo a tutte, lo dobbiamo a Maria, lo dobbiamo a tante giovani

Signora Presidente, signora Ministro, colleghe e colleghi, il tema dell'immagine della donna nei *media*, ma non solo, è stato già discusso in quest'Aula, e sono ormai moltissimi gli atti istituzionali di indirizzo che hanno cercato di imprimere una svolta alla deriva che è sotto gli occhi di tutti. Ricordo un documento del comitato TV e minori del 2004 e poi svariate risoluzioni del Parlamento europeo, sono già state citate, e anche del Consiglio, tutte volte a far sì che il ruolo della donna non venga ridotto nella pubblicità a una semplice icona di bellezza fisica e disponibilità sessuale, non invii messaggi di tipo discriminatorio, degradante e basati sul genere, non contenga elementi che possano indurre a violenze contro le donne e soprattutto non produca stereotipi di genere. tratta di un tema importante ed essenziale nell'educazione dei giovani, perché lo stereotipo inculcato fin da bambini è quello che poi crea divisioni in famiglia, nel lavoro, nel senso di appartenenza, determina già allora che cosa è possibile e che cosa non lo è. Credo che sia da lì che sostanzialmente ha origine il famoso tetto di cristallo, e questo noi dobbiamo assolutamente evitarlo. In alcune delle mozioni oggi in discussione sono giustamente citati la Costituzione e il Trattato di Lisbona. Ho richiamato velocemente tale elenco per vari motivi. Il primo è che questo argomento tocca il rapporto donne-*media* nella società moderna: un problema esiste, e l'abbiamo visto da tutti gli atti che sono usciti in tutto il mondo globalizzato, o almeno dove i mezzi di comunicazione di massa, e ormai anche la Rete, hanno raggiunto una diffusione anche capillare. Il secondo motivo è perché tale tema tocca molto da vicino, profondamente, il rapporto uomo-donna. Il terzo motivo è perché è evidente che la soluzione del problema non è facile e, seppur meritori, gli atti di indirizzo semplicemente non bastano. Credo che ci debba essere un'assunzione di responsabilità e quindi un conseguente cambio di rotta da parte di tutti i soggetti interessati: i *media*, che da parte loro devono darsi definitivamente un codice di autoregolamentazione e rispettarlo, magari anche sotto minaccia - perché no? - di qualche sanzione; le famiglie, che hanno il compito di educare i propri figli al rispetto di se stessi e degli altri, al rispetto della figura femminile e del ruolo fondamentale della donna nella società, e che non possono far finta di niente e sperare che altri facciano per loro questo lavoro; la scuola, che deve rafforzare questi insegnamenti; poi le donne, che devono avere maggiore coscienza delle proprie capacità, maggiore rispetto per la propria intelligenza, maggiore consapevolezza del ruolo fondamentale che hanno sempre avuto in ogni società, maggiore tenacia nel raggiungere gli obiettivi che si propongono senza cercare scorciatoie; ultimo, ma non ultimo, gli uomini,

e che più di noi - perché più di noi occupano ruoli dirigenziali - potrebbero fare scelte diverse di *marketing*, oppure, nel ruolo di consumatori, scelte diverse di acquisto di programmi o di riviste (è noto, infatti, che al momento vende molto di più un nudo in copertina di un paesaggio montano). Quello che, invece, assolutamente non deve accadere è che le donne si dividano su questi temi, perché al di là di legittime posizioni ideologiche, che comprendo, questa è una battaglia che dobbiamo fare e vincere tutti insieme, anche gli uomini.

Devo dire che le nostre due ministre Carfagna e Prestigiacomo tanto si sono adoperate e sono riuscite ad ottenere

collega Garavaglia, insieme al Ministro

ed avevamo la consapevolezza che, nel momento in cui si sarebbe affermato il merito, noi donne - come stiamo del resto facendo - non avremmo avuto più problemi.

per prima cosa come donne. Perché noi dobbiamo esserci senza rinunciare alle nostre caratteristiche, alle nostre peculiarità, al nostro essere donne: se per lavorare ed esserci dovessimo trasformarci in altrettanti maschietti credo che per la società, che è composta già da tanti di loro, il nostro apporto, le nostre peculiarità, la nostra creatività sarebbero alla fine inutili. Passo ora a parlare della nostra mozione, quella che insieme a tanti altri colleghi abbiamo firmato e che parla, in generale, dell'influenza

certi istituti fondamentali che sono nostri riacquistino il valore che avevano uscendo dall'influenza dei messaggi che passano liberamente dai *media*. quindi alla mia breve illustrazione. Insieme a molti colleghi ho sottoscritto la mozione che stiamo discutendo perché in tanti abbiamo avuto la chiara percezione di un profondo mutamento del ruolo che i *mass media* stanno avendo a livello sociale. Al suo nascere, la televisione - ma il discorso vale anche per il più recente mondo multimediale - ha aiutato la crescita sociale e civile con programmi di utilità, facendo conoscere agli italiani popoli e culture diverse, informando in maniera sobria e ragionata e contemporaneamente presentando l'Italia al mondo. Questa è la globalizzazione. Oggi si riscontra una prevalenza di messaggi surreali, magari veicolati attraverso *reality* che influenzano negativamente soprattutto il comportamento di nuove generazioni, alle quali suggeriscono scorciatoie pericolose per la realizzazione personale. Il nostro popolo, è noto, ha costruito la sua storia e la sua cultura intorno a valori tradizionali, sui quali poi si sono fondate le nostre istituzioni democratiche. Purtroppo, la percezione di questi valori si è modificata nel tempo ed è stata messa in discussione dai *media*, sempre meno attenti ai contenuti, e forse non del tutto consapevoli della vastità delle ricadute negative. Nella mentalità corrente è passata l'idea che quello che va bene nella finzione televisiva e multimediale sia lecito ed opportuno anche nella vita di ogni giorno. Molti non riescono più a distinguere tra realtà e finzione. Ci sono stati molti casi di cronaca in cui, di fronte a tragedie causate dall'alcol, dalla droga, dalla noia, dalla solitudine, dalle incertezze, ci siamo chiesti: ma come è potuto capitare questo? Basta accendere la televisione e ogni giorno l'interrogativo sorge spontaneo nella nostra mente. È ora di cominciare a dare risposte a domande che riguardano il senso profondo della vita e la felicità vera delle persone. I *mass media* hanno dimostrato il loro potenziale soprattutto nel modellare le nuove generazioni. Lo hanno fatto indebolendo l'azione della famiglia, della scuola e dell'associazionismo. Così oggi ci si comporta come viene dettato dalla televisione e instillato dalla pubblicità; purtroppo in molti casi questo avviene. Anche l'innata generosità dei giovani, non curata, si va spegnendo: quanti sono morti di freddo in questi ultimi tempi, si è fatta strada un'idea di vita fondata sul successo e sul denaro come obiettivi per una realizzazione che alla lunga si dimostra falsa e insoddisfacente sul piano personale e dannosa su quello sociale. Si sacrifica la centralità della famiglia, si perde spesso anche la propria libertà pur di ottenere quella felicità disegnata - ma non per essere modello - nei film e negli *spot* pubblicitari. Mi verrebbe da dire che il bene, che pure c'è, non fa notizia: non passando in televisione potrebbe rischiare di sparire del tutto. Anzi, rischia di far apparire coloro che fanno il bene come una sorta di eroi lontani, impossibili da imitare, quasi fossero persone sbagliate in questa società contemporanea. Una delle principali cause della situazione attuale è il linguaggio pubblicitario (di questo molte colleghe hanno parlato, e mi dispiace che abbiano parlato solo le colleghe: i colleghi forse non sentono il tema, o lo snobbano),

Oggi questo linguaggio sembra ruotare quasi esclusivamente intorno al corpo femminile, con un impatto devastante sulle nuove generazioni. Quasi sempre la donna nella pubblicità è rappresentata da modelli non solo offensivi dell'intelligenza, ma sostanzialmente falsi e inadeguati ad affrontare la realtà, se presi sul serio. Come parlamentari, ci sentiamo di suggerire al Governo di mettere un freno a questa situazione e di fare in modo che i *mass media* tornino a contribuire per ricreare quella univocità di messaggi che è necessaria, assieme a famiglia e scuola. C'è una grande emergenza educativa in Italia, come hanno sottolineato anche i vescovi, e sarebbe davvero assurdo se si mantenesse l'attuale piano di antagonismo tra quanto trasmesso nei *media* e quanto a fatica cercano di costruire le agenzie educative tradizionali. Chiediamo dunque di sostenere la scuola, investendo sulla formazione degli insegnanti e inserendo nei programmi contenuti formativi e civici. È importante far capire che il bene comune è alla portata di tutti. Un messaggio particolare, specie per i giovani, per esempio, può venire sottolineando gli sport a livello dilettantistico, dove emergono doti che sono utili alla vita (abbiamo ascoltato ieri da Valentina Vezzali che cosa significhi essere persona di sport). I mezzi di comunicazione possono concorrere ad educare e formare i giovani dando spazio ai buoni esempi e alle buone prassi. Infine, vorrei scrivere un grande «basta» allo sfruttamento dell'immagine femminile come strumento pubblicitario e consumistico. Nella mozione chiediamo ai *media* una rivalutazione delle specificità e un'immagine reale della donna, non più stereotipata o banalizzata: un recupero che farà guadagnare dignità a tutta la società.

c'è chi ha detto, anche in queste ore, che la mozione sulle donne e il sistema dei *media* non è poi così importante, che ci sono altri strumenti per affrontare un tema così delicato e quindi che questa mozione in realtà non sarebbe così significativa. Noi non siamo d'accordo: lo strumento della mozione è importante per definire come intendiamo questo rapporto e cosa intendiamo fare. C'è una premessa: nel rapporto donne-*media*, cosa intendiamo per le donne di oggi, e se i *media* rappresentano adeguatamente le donne di oggi. Noi, cara Ministro, colleghe e colleghi, signora Presidente, eravamo e siamo pronti ad una discussione seria su questo, e le mozioni da noi presentate lo testimoniano, come del resto quelle presentate da altre forze dell'opposizione.

Si nota in questa mozione, nonostante lo sforzo pur fatto, un certo imbarazzo a guardare in faccia i cambiamenti intervenuti nella vita delle donne di oggi, nel loro difficile equilibrio tra tanti aspetti che la caratterizzano. Questo imbarazzo scivola spesso in ipocrisia. Nelle mozioni Lauro e Aderenti - mi spiace dirlo - le donne di oggi non ci sono, non le abbiamo viste. Non c'è la loro determinazione, nonostante le difficoltà, a trovare lavoro, mantenerlo, avere servizi adeguati, vivere serenamente i loro rapporti, personali e familiari, ad essere riconosciute pienamente come persone: come persone irriducibili a qualsiasi ruolo, identità di altri o relazioni. È questa la vera rivoluzione questa la vera rivoluzione che ha attraversato le donne nei decenni passati, e che le grandi manifestazioni di febbraio ci hanno mostrato in modo straordinario. Noi donne - e vogliamo dirlo con pacatezza ma anche con orgoglio - non vogliamo tornare indietro ed essere spezzettate, divise per ruoli. Noi siamo tante cose perché siamo un'unica persona e non stereotipi o strumenti. È questa la vera rivoluzione dei diritti umani: le donne come fine e non come strumenti. Nella mozione n. 226, a prima firma Franco Vittoria troviamo scritto che «negli ultimi anni la condizione generale delle donne è regredita al punto tale che l'immagine prevalente che ne deriva è quella degradata ad un oggetto di sfruttamento sessuale da valutare soprattutto per la prestanza fisica e la giovane età». In quella a prima firma Bonino si legge che «tutte le rilevazioni e le ricerche svolte, anche in tempi recentissimi, confermano che la rappresentazione delle donne nei *media* italiani si focalizza su pochi insistenti stereotipi relativi al corpo, alla bellezza, alla sessualità, o alla donna come vittima di violenza, angelo del focolare, a scapito di rappresentazioni di donne capaci, competenti, variegate come età e condizione». In quella a prima firma Carlino, è scritto che «la rappresentazione sessista della donna trasmessa dai *media* e dalla pubblicità incide soprattutto sulle giovani generazioni. Lo mostrano i risultati delle ricerche che hanno analizzato i processi psicologici di oggettivazione e di auto-oggettivazione». Come ognuno di noi può vedere (e sono le poche righe che ho citato di queste mozioni) le questioni poste sono una sferzante critica al divario tra le donne di oggi e la loro rappresentazione mediatica: sferzante critica che parte dalla consapevolezza che visioni conservatrici del ruolo delle donne sono oggi tanto più dannose perché si tratta oggi di disconoscere donne che ormai anche gli ultimi dati ISTAT lo dimostrano - hanno un primato in rosa anche nello studio, nel rendimento scolastico, nella lettura e perfino nel teatro. già non vi appassionate troppo; se almeno non disturbate, magari è meglio. SERAFINI Anna Maria *(PD)*. Se non ora quando? Questo vuol dire: ma è possibile che ancora in tanti oggi si cerchi di arginare, disconoscere, non rispettare l'enorme cammino fatto dalle donne in questi decenni? Care colleghe e colleghi, cara Ministro, le ironie facili sulle donne del centrosinistra le abbiamo sentite anche in questi giorni da parte di esponenti del centrodestra. Qualche battuta

sui diritti delle donne, sulla loro dignità, sulle lotte per affermarli ogni giorno. *(Applausi dal Gruppo* *PD)*. No, cara Ministro, non le accettiamo! L'umiltà deve essere di tutti, ma in primo luogo di chi governa e se l'occupazione femminile è la più bassa, se le spese per le famiglie sono la metà della *media* europea, se l'immagine della donna è la più degradata, deve preoccupare tutti, ma in primo luogo voi. Ecco, cara Ministro: se possiamo sintetizzare come abbiamo vissuto noi le mozioni che la maggioranza ha presentato (lo dico sentendo anche le altre colleghe e colleghi) purtroppo in questo dibattito la maggioranza ha perso un'occasione. Questo dibattito è un'occasione mancata. Diciamo questo con molta chiarezza e determinazione. Non si può pensare di affrontare la vita di oggi delle donne, i loro diritti, la rivoluzione che le donne hanno compiuto nel secolo scorso e che prosegue oggi senza una visione avanzata e progressista dei loro diritti. Una visione conservatrice che le spezzetta e riconduce *ad unum*, a degli stereotipi, non potrà mai far avanzare le donne nella loro dignità e nella loro vita.

vorrei dire che ho ascoltato con grande attenzione e con grande interesse gli interventi delle colleghe e dei colleghi, che sicuramente hanno prodotto riflessioni e spunti che serviranno come contributo all'attività del Governo nel prosieguo della sua battaglia per la promozione, la difesa e la tutela dei diritti e della dignità della donna. allora qualche riflessione e farò anche qualche precisazione sull'attività che il Governo ha portato avanti in questi anni per contrastare stereotipi diffusi e per contrastare l'uso distorto dell'immagine femminile che ancora, purtroppo, è diffuso all'interno dei *media* e della pubblicità in generale. L'utilizzo dell'immagine femminile nei *media*,e in particolare nella pubblicità, e il ruolo donne nei settori della vita produttiva, sociale e lavorativa, l'acquisizione di poteri da parte delle donne (il cosiddetto *empowerment* femminile) vedono il Ministero per le pari opportunità impegnato costantemente in azioni positive finalizzate al superamento di ostacoli e di barriere che esistono e continuano a condizionare l'*humus* culturale. La pubblicità, in particolare, com'è stato più volte sottolineato, ha un peso enorme nella proposizione e nella diffusione di modelli culturali. Vengono veicolati purtroppo modelli pubblicitari che non corrispondono alla realtà, in cui, per fortuna, così come ricordato dalle tante colleghe intervenute, sono tante le donne che dirigono aziende, che dirigono uffici, donne laureate, donne impegnate in politica.

e ribadire) che «per raggiungere una parità sostanziale è necessario incidere essenzialmente sulla cultura diffusa: sulla concezione del ruolo della donna, sugli squilibri persistenti e capillari nelle relazioni tra i generi, su un'immagine consumistica che la riduce da soggetto ad oggetto. Per favorire il cammino verso una parità sostanziale, molto devono fare la scuola e i mezzi di comunicazione attraverso i valori che trasmettono». Il Capo dello Stato ha inoltre affermato che spetta in particolare alle donne «offrire validi modelli di comportamento. Non solo a quante hanno particolari funzioni e visibilità, ma a tutte le donne spetta, nella quotidianità della loro vita, il dovere di contrastare luoghi comuni, di esigere rispetto e considerazione». Occorre dunque esigere il rispetto della dignità delle donne in qualunque circostanza. Come riportato nel documento sulla rappresentazione della donna nei *media*, elaborato dal Comitato *media* e minori nel 2009, se le donne studiano, se lavorano, se vedono rispettati i loro diritti e la loro dignità di persone, tutto questo contribuisce a far definire quella società come realmente avanzata e sviluppata. Ricerche autorevoli hanno messo in luce come talvolta l'immagine della donna nella comunicazione televisiva e pubblicitaria non corrisponda in alcun modo alla realtà sociale, non rappresenti le donne in modo veritiero, dal momento che la stessa comunicazione appare sempre più connotata da un ammiccamento erotico e spesso volgare. Il Comitato nazionale di parità uomo-donna operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che da vent'anni promuove le azioni positive nel mondo del lavoro per l'acquisizione di poteri e di responsabilità da parte delle donne in tutti i settori del mondo del lavoro, nell'associarsi a quanto espresso dal Comitato *media* e minori, ha sollecitato tutte le emittenti televisive ha sollecitato tutte le emittenti televisive a prestare maggiore attenzione ai modi in cui vengono rappresentante le donne nei vari programmi di intrattenimento e in special modo nella pubblicità, nella convinzione che bisogna combattere quella cultura che facilita l'affermarsi di una distorta rappresentazione della figura femminile. *(Applausi dal Gruppo PdL).* La tutela dell'immagine della donna nei *media* rappresenta un tema all'attenzione dell'Unione europea: basti citare a questo proposito la comunicazione adottata nel 2006 dalla Commissione europea intitolata «Una tabella di marcia per la parità tra uomini e donne», che ha inteso attribuire ai mezzi di comunicazione un ruolo importante nella lotta contro gli stereotipi di genere, e la risoluzione del Parlamento europeo del 2008 concernente l'impatto del *marketing* e della pubblicità sulla parità tra uomini e donne, con la quale è stato richiesto agli Stati membri di intensificare gli sforzi affinché la pubblicità sia tesa alla valorizzazione della figura femminile e del ruolo delle donne nella società, invitandoli a provvedere con idonei mezzi affinché il *marketing* e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non diano luogo a discriminazioni dirette o indirette e non contengano elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne. Proprio aderendo alle linee tracciate dalla Commissione europea, ho inteso siglare il 26 gennaio scorso un protocollo d'intesa con l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria che dal 1996 opera in Italia con lo scopo di affermare una comunicazione commerciale sempre più onesta, veritiera e corretta, anche attraverso la rigorosa applicazione del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. Il protocollo è finalizzato a rendere più efficace la collaborazione nel controllo e nel ritiro di pubblicità che sviliscano l'immagine della donna, con raffigurazioni o scene offensive e volgari o che sia apertamente sessista. In particolare, attraverso la stipula del citato protocollo, il Ministero per le pari opportunità e l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria si impegnano a collaborare per fare in modo che gli operatori di pubblicità e i loro utenti adottino modelli di comunicazione commerciale che non contengano immagini che non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne; che tutelino la dignità della donna; che rispettino il principio di pari opportunità; che diffondano valori positivi sulla figura femminile; che siano attenti alla rappresentazione dei generi e rispettosi delle identità di uomini e donne, coerenti con l'evoluzione dei ruoli nella società e che evitino il ricorso a stereotipi di genere. Attraverso tale protocollo, il Ministero per le pari opportunità potrà chiedere, come già avvenuto in molte occasioni, il ritiro di una pubblicità in tempo reale, comunque entro 48 ore, riuscendo a monitorare la comunicazione pubblicitaria nella sua quasi totale interezza, dal momento che l'Istituto

Quanto all'imminente stipula del Contratto di servizio 2010-2012 con la RAI, occorre rimarcare il suo forte contenuto innovativo sul tema di una diversa rappresentazione del ruolo della donna nella società, atteso che il Ministero dello sviluppo economico e la RAI hanno recepito pressoché integralmente le proposte formulate dal comitato «Donne e *media*» e dal comitato «Pari o dispare» nella fase di stesura finale del testo. In tale quadro, più in particolare, il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI hanno integralmente recepito la proposta della Commissione parlamentare di vigilanza che richiede alla RAI di realizzare un «monitoraggio...che consenta di verificare il rispetto delle pari opportunità, nonché la corretta rappresentazione della dignità della persona nella programmazione complessiva, con particolare riferimento alla distorta rappresentazione della figura femminile, e di promuoverne un'immagine reale e non stereotipata. I *report* dovranno essere trasmessi al Ministero, all'Autorità, e alla Commissione parlamentare». Per quanto concerne invece la valorizzazione del ruolo della donna nei campi artistico, culturale, scientifico e politico a cui si fa riferimento in alcune mozioni, vorrei sottolineare che in Italia il numero di donne che persegue una carriera scientifica è cresciuto notevolmente negli ultimi vent'anni. Secondo il Rapporto del 2009 della Commissione europea «*She Figures* - Statistiche e indicatori sulla parità di genere nella scienza», le donne rappresentano il 33 per cento dei ricercatori italiani, dunque una media superiore a quella europea che si attesta, invece, al 30 L'interesse delle istituzioni si concentra sull'accesso e sulla partecipazione delle donne, specialmente di media età, alla formazione nei settori scientifico e tecnologico, in considerazione dell'attuale quadro di un'economia sempre più basata sulla conoscenza. Occorre quindi compiere ogni sforzo per superare situazioni di disparità di genere in tali settori. Consapevole di questo, vorrei segnalare due importanti progetti coordinati dal Ministero per le pari opportunità: il progetto «*Practising Gender Equality in Science*», che ha avuto il merito di mettere a sistema le buone pratiche nel settore della ricerca scientifica e si è concluso nel 2009 con la pubblicazione delle «Linee guida per la parità di genere nelle scienze», il progetto «*Women Careers Hitting the Target*», che si concluderà invece a luglio 2011 e si occupa di monitorare, dirigere e analizzare la diversità di genere nel mondo della ricerca pubblica universitaria. Entrambi i progetti sono stati coofinanziati dall'Unione europea. Inoltre, considerato che l'avanzamento delle donne nelle carriere scientifiche rappresenta un settore cruciale per il futuro sviluppo dell'Europa, nel settembre 2010 ho siglato, insieme al Ministro dell'istruzione, un protocollo d'intesa finalizzato a elaborare misure concrete per conseguire la parità di genere nella scienza, combattere la sottorappresentanza delle donne nei settori scientifici, favorire l'avanzamento delle carriere delle donne, migliorare la presenza delle donne nel mercato del lavoro nel settore scientifico e, in particolare, nei posti decisionali. Ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 36 della Dichiarazione di Pechino del 1995, dalla Comunicazione «*Women and Science*» adottata nel 1999 dalla Commissione europea, nonché dalle raccomandazioni agli Stati membri dell'Unione europea contenute nel Position Paper «*Gender and Research Beyond 2009*», adottate il 24 novembre 2009 dal Gruppo di Helsinki su Donne e Scienza, in cui si esprime un chiaro impegno a mobilitare le donne per contribuire in maniera essenziale al completamento della *European Research Area*. In merito alla valorizzazione del lavoro delle donne nei campi artistico e culturale, segnalo che, come riferito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel campo delle Accademie di belle arti viene pienamente rispettata la parità dei diritti tra uomini e donne per l'accesso a cariche di responsabilità, in quanto tutte le nomine degli organi di governo avvengono sulla base di un sistema elettivo che, direttamente o indirettamente, coinvolge l'intero corpo docente. Nel corso dell'ultima sessione sulla condizione delle donne presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, tenutasi a New York lo scorso 22 febbraio, ho avuto modo di illustrare le iniziative poste in essere dal Governo italiano al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e delle pari opportunità tra uomini e donne, specie per quanto attiene all'ambito occupazionale. Naturalmente, l'impegno in questa direzione non deve sminuire il fondamentale ruolo della donna

dicevo, l'impegno in questa direzione non deve sminuire il fondamentale ruolo della donna all'interno della famiglia, ed alla conciliazione di questo ruolo con gli impegni lavorativi sono protesi tutti i nostri sforzi, da ultimo culminati nell'importante accordo siglato il 7 marzo con le parti sociali per inserire nella contrattazione collettiva nuove regole *family friendly,* quindi favorevoli alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne. a questo scopo che 40 milioni di euro sono stati stanziati dal Ministero per le pari opportunità per misure che le Regioni stanno già mettendo in campo a favore delle donne che lavorano. Possono aiutare sicuramente alla costruzione di un'immagine diversa della donna anche interventi legislativi, come quello sulle quota rosa nei consigli di amministrazione delle aziende, che stamattina ha avuto un via libera importante. Per questo vorrei ringraziare tutte le senatrici impegnate per l'ottimo lavoro svolto, che ha portato a costruire una normativa sicuramente equilibrata ed efficace.

soltanto per rinnovare la richiesta di avere notizie certe circa i tempi per la presentazione del bilancio interno del nostro Senato. Tutti gli anni ce ne accorgiamo sempre un po' avanti si è poi posti di fronte alla necessità di preparare documenti che affrontino nel dettaglio un documento corposo, quanto prima questo viene reso noto

una forchetta tra lo 0,01 e lo 0,05, che oltre a ridurre la speculazione, potrebbe generare introiti per 250-300 miliardi di euro l'anno da destinare a nuovi posti di lavoro e ad investimenti nelle infrastrutture per cercare di dare risposte alla crisi generata dai banchieri. Voglio ricordare ai colleghi che l'Italia dei Valori ha depositato da tempo in Senato a mia prima firma una proposta di legge per introdurre la Tobin *tax*, in armonia con le decisioni assunte dall'Europa, anche per calmierare quelle quotidiane speculazioni di una ristretta oligarchia di banchieri collusi con autorità vigilanti che predicano bene e razzolano male, e che decidono in segreto i prezzi dei *futures* sul petrolio, sul grano, sulla soia e su quelle materie prime i cui aumenti hanno generato in Nord Africa la rivolta di popolo e di giovani senza futuro, definita «la guerra del pane». Anche perché, in assenza di decisioni, che il G20 continua a rinviare, questi banchieri continuano a giocare con i derivati, generando gigantesche piramidi finanziarie con strumenti OTC (*Over the Counter*) scambiati fuori dai mercati regolamentati per centinaia di milioni di dollari, su cui fondano i loro profitti e le loro *stock option*. Per i *bankster* «il tempo del rimorso», dopo i disastri che hanno provocato, non è finito. Bob Diamond, presidente e amministratore delegato della Barclays Bank, ha spazzato via ogni residuo rimorso per le responsabilità che banche e banchieri hanno avuto nella crisi. Ora nella City di Londra è tornato il tempo dell'avidità,

devono fare presto regole nuove e sanzioni dure, per evitare future catastrofi che incombono sulla pelle dei popoli e della sovranità degli Stati.

il ministro Bondi ha ricevuto 100 autori della cinematografia italiana che hanno lanciato un appello in difesa di Cinecittà e dell'Istituto Luce. Luce. È un argomento sicuramente importante. Forse qualcuno non ricorda che Cinecittà è stato ed è ancora nel mondo della cinematografia italiana ed internazionale un punto di riferimento importante. Ancora prima di Hollywood, Cinecittà è stato un impegno concreto del grande cinema realista italiano. Quindi, rivolgo un appello affinché il Presidente del Senato intervenga nei riguardi di tutti gli enti preposti alla salvaguardia non solo dei posti di lavoro, ma di un ente, come l'Istituto Luce, che raccoglie la storia della cinematografia italiana e mondiale.

in quest'Aula ci ricorda sempre il grande tema della finanza, delle intermediazioni e delle speculazioni finanziarie, che poi hanno avuto e continuano ad avere pesanti ricadute sull'economia reale.

- negli anni delle lusinghe della grande ingegneria finanziaria del sistema anglosassone non ha risposto in modo positivo, mantenendosi invece ancorato a meriti di credito storicamente più consolidati

che però oggi rischiano di appesantire anche noi. Vorrei lasciare all'ufficialità di questa Assemblea una riflessione, che mi auguro anche altri possano condividere, nel difendere il sistema bancario italiano dalla scure di Basilea 3 in tutti i modi. Recentemente il Senato, approvando il decreto milleproroghe, ha

Presidente, vorrei associarmi all'appello del collega Gramazio sulla vicenda di Cinecittà, ma ci tenevo anche a ricordare che quest'Aula non si può accorgere delle cose che esistono solo a un certo punto, quando già sono scoppiate, senatore Gramazio, e che soprattutto... GRAMAZIO *(PdL)*.

Tra l'altro, il ministro Bondi, che ieri ha ricevuto i 100 autori - non so se li ha ricevuti al Ministero, perché si dice che non ci vada da molti mesi deve smetterla con questa pantomima, di cui c'è stata una coda sui giornali dei giorni scorsi: se non ce la fa, come è evidente, se ne vada subito, e non aspetti le calende greche. Vorrei solo ricordare a quest'Assemblea - mi dispiace che non ci sono alcuni colleghi della Commissione bilancio, ma ne ho parlato già nelle dichiarazioni di voto - che noi presentammo tutta una serie di emendamenti sul Fondo unico per lo spettacolo, il noto FUS, che è stato ridotto e portato da circa 500 milioni a 250 milioni di euro; che abbiamo votato contro quella farsa che restituiva pochi milioni di euro alle fondazioni

il problema dell'Istituto Luce, del Centro di cinematografia, di un pezzo di cultura che ha fatto grande questo Paese e che affonda le proprie radici non nella mia storia, senatore Gramazio, ma nella sua

dalla vostra disattenzione. Quindi sono contento che oggi si arrivi, a cose fatte, a scoprire che non ci sono i fondi. Potevate farlo prima! molto breve, ma non potevo non esprimere anch'io la mia solidarietà al collega Gramazio, con il quale, come sapete, ho una relazione particolare in quest'Aula. Il collega Gramazio ha fatto una citazione colta:

Tagliare un'industria significa avere cattive politiche industriali, significa essere mercatisti. Questo è Tremonti: un mercatista. Rispetto a Roma, ha tagliato a Cinecittà, non dimenticandosi però, come il sindaco di Roma, forse dopo gli ultimi «Stati generali», di cambiare il responsabile di «Musica per Roma», dopo il bel lavoro fatto prima da Borgna, mettendoci un suo uomo, e senza dimenticarsi le poltrone... GRAMAZIO *(PdL)*.